la partecipazione dei privati alle fondazioni lirico-sinfoniche. Non si è però ricordato abbastanza come i Governi di centrosinistra avessero previsto una dotazione finanziaria significativa per lo sgravio fiscale, che è stata poi cancellata nel 2001 dal ministro Tremonti.

che detto trasferimento potrà essere ridotto soltanto in presenza di un contemporaneo ed adeguato apporto finanziario di parte privata. Da ciò scaturisce l'importanza di questo emendamento che chiedo di votare.

**Il Senato non approva**.

in sostanza si vorrebbe, a garanzia della qualità produttiva, perlomeno il mantenimento dell'attuale consistenza organica dei complessi stabili. Pensate se, a stagioni già avviate,

chiusa, rigida rispetto ad una logica di maggiore trasparenza, di buona e corretta gestione e amministrazione, di effettiva responsabilità, produttività e qualità.

l'indice di produttività, i livelli qualitativi della produzione svolta, il numero degli spettatori, il numero delle coproduzioni (che poi è un punto importantissimo rispetto al futuro delle fondazioni

positiva voluta dal Governo di centrosinistra, introdotta dal ministro Rutelli e poi, dopo vari ripensamenti, confermata dell'attuale

di buonsenso, che effettivamente coglierebbe l'obiettivo, il centrodestra si tira indietro. Si evince con forza e chiarezza quali sono le reali le reali volontà di questa maggioranza e di questo Governo: ovviamente non sono quelle di creare le condizioni affinché gli enti lirico-sinfonici possano negli anni futuri funzionare bene ed arricchire e valorizzare il patrimonio

la Lega votare contro la condivisione normativa da parte delle Regioni, vediamo ora il centrodestra, che dovrebbe essere spinto naturalmente ed ideologicamente verso l'allargamento ai privati, ancora una volta parlare in un modo ed agire esattamente nel modo

ci aspetteremmo una grande unità, visto che sul punto di Santa Cecilia si è raggiunta prima una identità di intenti, in quanto non sfugge a nessuno che si tratta di uno dei fiori all'occhiello dell'Italia nel mondo. È noto e non c'è bisogno che lo aggiunga. Dunque, ci auguriamo che questo emendamento 1.0.300,

attiriamo l'attenzione su tutte le fondazioni; è altrettanto chiaro che condivido assolutamente l'impostazione che il mio Gruppo ha dato.

seria rispetto alla immagine che questa istituzione offre nel Paese e del Paese se sia il caso che con questo provvedimento mettiamo in difficoltà proprio uno di quei punti di eccellenza che fanno l'identità del nostro Paese all'estero.

però è una fase importante, colleghi della maggioranza, perché un Governo che, per quanto riguarda le politiche culturali, accentra senza destinare non si capisce che politica abbia, signor Ministro. È chiaro che il Governo può decidere di dare corso alla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche secondo un'indicazione che magari è in linea con la posizione di alcune formazioni politiche della maggioranza - penso alla Lega - le quali immaginano che anziché un centralismo romano si debba dar corso alle capacità e potenzialità del territorio. Come è emerso finora e anche alla luce degli interventi del collega Marcucci, che sottoscrivo, ciò è stato respinto. L'opposizione ed il Partito Democratico hanno presentato degli emendamenti che propongono un meccanismo innovativo,

cioè un credito d'imposta che permetta investimenti virtuosi nel settore. La maggioranza ha respinto anche questa posizione. Parimenti, è stata avanzata la proposta di favorire le erogazioni liberali, cioè creare dei meccanismi di incentivo per coloro che vogliono finanziare un settore così particolare della nostra cultura.

e sappiamo bene come, in particolare, le fondazioni lirico-sinfoniche ricevano percentualmente risorse molto maggiori - se si vuole anche sproporzionate - rispetto agli altri comparti dello spettacolo a causa dei costi molto particolari di questo settore.

l'impostazione di credito d'imposta e l'impostazione delle erogazioni liberali, ci si immagina che scegliate dei meccanismi di merito

culturali del nostro Paese. Poco fa il collega Vita si è riferito all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che certamente merita un'attenzione non meno specifica. Come fate, dopo avere bocciato tutte le opzioni alternative, anche a bocciare magari, signor Ministro, anche con una previsione di disponibilità inferiore a quella che viene proposta con questo emendamento - il luogo di massima eccellenza della cultura musicale italiana

È evidente dal complesso di queste proposte emendative, che vengono rigettate una dopo l'altra, che c'è la volontà di blindare questo testo, ma senza un costrutto ed una logica e senza dare un futuro alla cultura italiana. Questo è il momento, signora Presidente, nel quale credo forse il Ministro dovrebbe dire quali sono le priorità, perché dire semplicemente no a tutti gli orientamenti alternativi per far vivere queste grandi istituzioni significa semplicemente condannarle a morire.

due considerazioni. Innanzitutto, sul fatto che occorrono maggiori energie finanziarie per il settore degli enti lirici siamo tutti d'accordo,

indipendentemente dalla situazione economica di ognuno, chiedono un maggiore esborso da parte dello Stato come finanziamento; mi sembra quasi una distribuzione a pioggia, indipendentemente dalla

pensare che non si vada ad un riordino per rendere più virtuosi molti degli enti lirici del Paese significa vivere in un altro mondo. Questo si chiede, non altro. Lo dicevo ieri: dobbiamo ricordare a tutti che quando si spendono soldi dello Stato sono soldi che i cittadini italiani versano con le tasse; bisogna essere particolarmente oculati nella spesa, perché non vengono dal cielo: sono i sacrifici che con le tasse fanno i cittadini italiani, specie gli operai, specie gli ultimi, quindi, quando si spendono, si devono spendere con oculatezza. Non si può pensare che un ente lirico più alza il sipario più spende, perché ogni volta ci sono costi aggiuntivi. Dovrebbe essere il contrario, come avviene nel resto del mondo: più si alza il sipario più si guadagna. In Italia è il contrario: vogliamo affrontarlo? Vogliamo verificarlo?

sugli sprechi che voi stessi avete favorito e determinato, quando ne avete avuto l'occasione. Ciò detto, in questo momento, ed è al Ministro che mi sono rivolto, voi non potete scartare contemporaneamente tutti i meccanismi di responsabilizzazione del territorio,

almeno simbolicamente uno degli emendamenti. Sono d'accordo con lei, è sbagliato dire che attribuiamo 10 milioni di euro dal Teatro al Teatro alla Scala ed è per questo che sono intervenuto a proposito dell'emendamento per il Teatro alla Scala: almeno il Governo dichiari che individua l'una o l'altra di queste fondazioni, per proprie valutazioni, poiché spetta al Governo e non all'"autodeterminazione" delle realtà territoriali alle quali voi vi state orientando ad attribuire il potere. Oggi il Governo, nel corso di questa discussione, dica almeno alla Scala di Milano merita una particolare attenzione. Non dica che gli si debbano attribuire 10 milioni di euro, come propone questo emendamento, ma dia un segno di attenzione specifico. Quindi, la mia domanda rivolta al collega Asciutti è: quale ordine del giorno, di grazia, dovrei presentare, quello che chiede più soldi per la lirica? Contraddirei esattamente quanto lei mi chiede, cioè dei criteri

del Teatro del Maggio musicale fiorentino è nota in tutto il mondo, e anche in quest'Aula credo che nessun possa avere il coraggio di negarlo. Negli anni, il Maggio musicale fiorentino ha conquistato il mondo, ha portato Firenze e l'Italia in tanti Paesi; è anche evidente a tutti che negli ultimi anni anche tale manifestazione è stata penalizzata dai tagli al FUS, che sono cresciuti nel tempo.

Devo anche ricordare che è in corso un investimento notevole per il nuovo auditorium per la musica di Firenze, con un investimento di oltre 100 milioni di euro di euro tra Stato, Regione Toscana ed enti locali, però si continua a tagliare le risorse e soprattutto, con questo decreto, si impediscono le assunzioni che consentirebbero di mantenere alta la qualità, ad esempio, dell'orchestra. Per tutti i teatri importanti chiediamo un contributo supplementare almeno in via eccezionale; con questo emendamento

E non per campanilismo, colleghi, ma perché dobbiamo sapere che più scade la qualità culturale delle singole istituzioni,

sede di fondazione lirico-sinfonica ha il valore di richiamare la discussione su un punto, che è quello che molto opportunamente ha ricordato il senatore Rutelli, e cioè che in presenza dei

provare a dire già per decreto quali delle fondazioni lirico-sinfoniche nel nostro Paese devono chiudere. Infatti, molte di quelle che si trovano in situazioni economico-finanziarie complesse - ed il Teatro comunale e la Fondazione lirico-sinfonica di Bologna sono tra queste - hanno in corso processi di ristrutturazione del debito e di riorganizzazione della gestione; ad esempio, a Bologna, nel corso dell'ultimo anno ha ha dimezzato il proprio *deficit* operando una serie di scelte di maggiore efficienza nella gestione e favorendo un percorso di partecipazione degli enti locali, delle istituzioni del territorio e della cittadinanza associata a sostegno del Teatro. È stato ristrutturato anche lo stato patrimoniale del Teatro, ma in presenza del permanere dei tagli al Fondo unico e data l'assoluta insufficienza delle misure di contenimento del solo costo del lavoro previste dal decreto, non si riuscirà a portare a termine alcun processo di ristrutturazione in quanto già a partire dal prossimo anno la conferma dei tagli porterebbe al *default* del Teatro. Quindi delle due l'una: si dia ai teatri l'autonomia di gestione loro necessaria per definire il proprio percorso di riorganizzazione e ristrutturazione e di scelta di fonti alternative di finanziamento,

dopo la collega Ghedini, che ha parlato del Teatro di Bologna, io, che sono di Genova, parlerò del Teatro di Genova.

un momento del mio intervento, ma ci è chiaro, che questi emendamenti siamo stati costretti a presentarli per porre l'attenzione sul fatto che all'interno di questo provvedimento - come ricordava giustamente il senatore Rutelli

di fondo: complessivamente la riforma non regge e, se così intendete proseguire, ciascuno per la propria città cercherà di trovare delle modalità per non far chiudere istituzioni culturali importantissime. Peraltro, parlando del Teatro Carlo Felice,

Di ciò parlerò in un successivo emendamento. Dico questo perché immaginavo che in una revisione complessiva degli enti lirici, rivedendo quanto è successo negli anni, si

la nostra contrarietà al provvedimento nel suo complesso.

in quest'ambito. Come i colleghi hanno avuto modo di ascoltare, si tratta di un gruppo di emendamenti che hanno anche un valore simbolico, e soprattutto, ci danno l'opportunità di parlare di ognuna delle 14 fondazioni del nostro Paese. Infatti, siamo convinti - vogliamo ribadirlo - che ogni teatro lirico abbia una sua specificità,

Dall'altra parte, con questi emendamenti vorremmo stigmatizzare ancora una volta

il Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, vorrei ricordare che si tratta di un teatro che ha valenza regionale, visto che è l'unico teatro lirico nella Regione Friuli-Venezia Giulia, e che sempre più sta diventando anche un punto di riferimento in un'area più vasta, transfrontaliera, visto che la musica non ha confini;

perché riteniamo che si dovrebbero premiare le fondazioni virtuose, quelle che in questi anni si sono sforzate per ripianare i debiti. Tra queste c'è anche il Teatro lirico Giuseppe Verdi, che negli ultimi due anni

abbia il più basso contributo privato. Riteniamo che tali sforzi, nel caso specifico operati dal sovrintendente insieme agli altri soggetti coinvolti nella gestione del teatro, andrebbero premiati. Si tratta comunque di un'attività ricca di produzione non solamente nei settori della lirica e del balletto, ma anche in quello concertistico

che uno dei settori più importanti che costituisce l'identità culturale e civile del nostro Paese è proprio quello della cultura, dei beni artistici, della lirica. Le fondazioni sono il nostro fiore all'occhiello. Eppure, anziché trovarci davanti ad una strategia di crescita e di rilancio, ci troviamo dinanzi ad una logica che si adagia esclusivamente sui tagli.

Il Governo e la maggioranza devono assumersi le loro responsabilità ed essere consapevoli fino in fondo delle scelte che vanno ad adottare in un settore

e temi di altissima qualità nel nostro Paese, che prescindono dalle maggioranze e che costituiscono un valore per tutti, per il patrimonio culturale, artistico e civile del nostro Paese.

Democratico ha presentato proprie proposte e ha condiviso, con i colleghi della Commissione di merito, atti di indirizzo della riforma stessa. Che i privati dovessero entrare di più nella vita degli enti lirici era per noi atto ineludibile, tanto da chiedere la defiscalizzazione dei contributi dei privati. Che bisognasse combattere gli sprechi significa per noi aprire una porta già spalancata: per questo le proposte di coordinamento delle fondazioni nella programmazione. Ma la domanda, signor Ministro, che le abbiamo rivolto anche in Commissione è: il Governo vuole espandere o restringere la forza e il prestigio degli enti lirici? Vuole consolidare l'importanza dell'opera nella cultura, non solo italiana? O vuole restringere il settore, ritenuto, tranne qualche eccezione, un peso a partire da un lavoro creativo poco incline, oltre una certa misura, a semplificazioni? Tale impressione è rafforzata laddove si pongano in alternativa superamento della crisi e investimento sulla cultura. C'è chi non li pone in alternativa, all'opposto li pone in una relazione strettissima. Proprio in questi giorni un suo collega, il ministro della cultura il ministro della cultura tedesco, Neumann, ha affermato: «Nonostante la crisi, Berlino non ha fatto tagli alla cultura. Anzi, il bilancio federale è aumentato per la quinta volta consecutiva nel 2010. È proprio in tempi di crisi che si deve lottare per non fare tagli alla cultura, perché è il valore e il fondamento che dobbiamo mantenere». *(Applausi dal Gruppo PD).* In riferimento agli enti lirici lo stesso Neumann afferma: «Pensare all'Italia significa pensare alla grande cultura».

più seri lo dimostrano), hanno un costo oggettivo che il loro riscontro economico non compenserà mai. In alcuni atteggiamenti offensivi della dignità della cultura sembra di rivedere gli attacchi continui, martellanti, che certa stampa quotidianamente sferra contro l'autorevolezza della politica, delle istituzioni. Non manca giorno che il populismo sguaiato attacchi il lavoro parlamentare, il nostro *status*, la dignità di ognuno di noi. dunque, ai presidenti Schifani e Fini: non soffrite anche voi dell'offesa che ci viene recata ogni giorno? È vero che spesso è miserevole e miserabile il punto da cui parte la critica, ma questa miseria si rovescia su ognuno di noi. La politica viene irrisa, risulta spreco anche in quanto attività intellettuale. Veniamo denigrati anche per questo e per il fatto che in questo caso il pensare, il prendere decisioni è proprio, democraticamente, di molti provenienti da ceti sociali non forti. Non disturba proprio questo? Stiamo attenti al populismo, da qualsiasi parte provenga. C'è chi dice, signor Ministro (c'è anche in un sito del centrodestra): perché finanziare l'opera, gli enti lirici, cultura alta a cui accedono i ricchi, con i soldi di tutti e, quindi, anche degli operai? Dopo Eco, pensavamo fosse una questione risolta. Questo modo di porre la questione è sbagliato per due motivi: il primo riguarda proprio l'ambito culturale e l'accesso alla cultura. L'elitarismo, lo snobismo, sono senza dubbio vizi capitali in cui rimangono imprigionati i veri poveri di spirito, quali siano il loro reddito e le loro frequentazioni culturali. Ma qui si tratta di altro: si contrappone all'elitarismo una sorta di populismo anticulturale. Per sconfiggere il populismo anticulturale, che spesso è il filo conduttore di alcuni commenti sull'attività degli enti lirici, occorre abbandonare l'identificazione della cultura con i grandi numeri o ritenere che solo i piccoli numeri costituiscono la vera cultura. È che spesso la cultura *tout court* viene identificata con lo spreco o qualcosa che riguarda solo i ceti colti o benestanti. Spesso è così. Senza dubbio non dovrebbe essere solo così, ma non si può fuoriuscire della ristrettezza del numero di chi accede alla cultura indebolendo la cultura medesima. Ad esempio, la maggiore risposta al populismo e all'espansione del settore degli enti lirici non può che essere, come premesso, il far propria con convinzione l'importanza di una migliore educazione musicale dei ragazzi, il cui livello questo è il punto da prendere in seria considerazione. La seconda questione, a cui molte colleghe e colleghi hanno fatto riferimento (da ultimo il senatore Procacci), riguarda l'identità culturale e come questa influenzi la possibilità di espansione di un moderno turismo.

Perché i cittadini di grandi Paesi, di antiche civiltà in rapidissimo sviluppo dovrebbero preferire l'Italia? Perché cittadini europei, americani, giapponesi dovrebbero scegliere il nostro Paese? Pensiamo che sia sufficiente il patrimonio culturale italiano, compresa l'opera, o che sia indifferente questo patrimonio? Ecco, l'emendamento che io ed altre colleghe e colleghi presentiamo riguarda il Teatro Massimo di Palermo. Ministro Bondi, lei dice che il provvedimento vuole premiare i virtuosi. Ebbene, il Teatro Massimo ha risanato il suo bilancio: ora ha bisogno di sviluppare tutte le sue potenzialità, al servizio di Palermo, della Sicilia e del Paese.

Presidente, signor Ministro, intervengo su questo emendamento, e relativo al Teatro dell'Opera di Roma, perché questo argomento è, in un certo senso, sintesi e metafora di tutto quello di cui stiamo parlando. Ha detto già molto bene

Il Teatro dell'Opera di Roma aveva ricevuto, con il sovrintendente di allora Ernani, rimosso poi dal sindaco Alemanno, un encomio da parte della Corte dei conti, perché esiste anche una classifica dei migliori bilanci. Dunque, il bilancio fu risanato e rispetto alla stagione che il senatore Rutelli prima ha ricordato tante cose erano cambiate: tra le altre, un direttore artistico tra i più giovani del nostro Paese e molto stimato a livello internazionale, Nicola Sani, stava aprendo il teatro ad un pubblico giovanile e anche a un repertorio diverso. tutti gli ingredienti, anche la qualità storica di Carla Fracci, che era a capo del corpo di danza, per rilanciare l'Opera di Roma che, purtroppo, a differenza di altri teatri di città che sono state qui ricordate, così importante, chissà come mai storicamente è meno inserito nel tessuto culturale della Capitale di quanto lo siano appunto altri stabili in città magari più piccole. E, dunque, questo sforzo davvero straordinario che tutti quanti, da varie parti politiche, cercammo di accompagnare con rispetto, anche in attesa - se ne parlava già allora - dell'arrivo del maestro Muti, è stato, signor Ministro, interrotto interrotto bruscamente con un sorta di commissariamento deciso a tavolino per motivi che non saprei identificare, perché da allora i conti economici non sono certo migliorati,

che non ha avuto ancora la possibilità e l'opportunità di conoscere gli stessi lavoratori. Lei ricorda chi è il nuovo direttore del personale, vice sindaco Cutrufo? Dovrebbe saperlo, lei è a capo dell'amministrazione. Glielo dico io: si chiama Massimo Salza, e anche lui non è stato conosciuto né all'interno né all'esterno. E il direttore generale, lo sa chi è? È il dottor Antonio Liguori, glielo dico io, nemmeno lui conosciuto né all'interno né all'esterno. Molta riservatezza da parte di questi nuovi dirigenti del Teatro dell'Opera che hanno preso il posto di alcune figure storiche

se ci sono dei premi economici (con questo emendamento, signor Ministro, vogliamo venire incontro persino al Governo), diciamo un contributo in più al Teatro dell'Opera di Roma. Ora è diretto da persone assai più vicine ai vostri orientamenti, benissimo, ma diamo lo stesso questo piccolo contributo perché la città di Roma

A questo emendamento che ha avuto uno dei pochi voti unitari voglio riferirmi perché nei punti *e)*, *f)* e *g)* del comma 1-*bis* dava qualche spazio di intervento e di ulteriore riflessione in questa materia. A tale riguardo, ministro Bondi e senatore Asciutti, qualche profonda autocritica va fatta, perché il tempo di intervenire c'era perché su misure strutturali per intervenire nella crisi che si stava addensando sulle fondazioni liriche già lavorammo insieme nella precedente legislatura con il disegno di legge del senatore Fontana. In ogni modo, la riflessione unitaria del Senato si è concentrata su tre punti: la necessità di prevedere valorizzazioni specifiche dei punti di eccellenza regionali; la necessità di esaltare quelle fondazioni che hanno un'offerta complessiva di lirica, di balletto, di musica sinfonica e attività produttive locali;

rilevanti. Riferendomi a questa selezione di possibili interventi noi crediamo - io credo - che si debba considerare - la cifra è simbolica, ma il simbolismo vale un necessario e specifico intervento per il Teatro Regio di Torino. Io credo che sia motivo d'orgoglio per tutti i senatori piemontesi, non importa se di maggioranza o di opposizione, sapere che il Teatro Regio di Torino non è nei parametri del ministro Bondi. Il Teatro Regio di Torino non riceve dal FUS il 60 per cento, ma, su un bilancio di 40 milioni di euro,

quale che sia il loro futuro colore, a sopperire sostanzialmente alle esigenze di un teatro che ha eccellenze internazionali e un profondo radicamento sul territorio e autosostentamento a livello regionale. Il Teatro Regio di Torino è da molto tempo in attivo;

Il Teatro Regio di Torino, il 17 marzo 2011, con i "Vespri siciliani", alla presenza del Presidente della Repubblica, inaugurerà tutte le manifestazioni del 150º anniversario dell'Unità d'Italia. Credo che almeno i senatori piemontesi, in forza della storia di questo teatro, della sua eccellente conduzione economica e del suo ruolo internazionale e nazionale, possano avere un attimo di considerazione libera e di prospettiva.

contraddizioni fra i principi generali posti a sostegno del decreto-legge in esame e le norme specifiche che il Governo vorrebbe introdurre in maniera molto limitata e negativa a sostegno delle attività liriche,

ma credo che ci scontreremmo contro una chiusura assoluta della Lega che, da una parte, parla di federalismo e di autonomia gestionale e finanziaria e, dall'altra, quando si trova a Roma,

Poco fa la senatrice Serafini ha ricordato le affermazioni di un ministro tedesco, di un Governo che fa la manovra più dura di tutta l'Europa, 80 miliardi di euro. Quindi, collega Asciutti, non ci dimentichiamo che siamo in crisi. Noi apparteniamo ad un *club* di Paesi fortunati, quelli europei, che tuttavia devono attraversare una grave crisi; però sulla cultura

per altri alzare il sipario a data prefissata è garantito; a Verona non è detto che si riescano a fare tutte le rappresentazioni a causa del fatto, che il tetto è il cielo. Quando è stellato potrà vedere che meraviglia di spettacolo e comunque all'inizio, già con le fiammelle, è veramente emozionante. Credo che tutti gli italiani abbiano avuto la possibilità di vederlo qualche sabato fa alla televisione. Quest'anno manterrà per tutta la stagione le scenografie e la regia di Zeffirelli, un nome che basta pronunciarlo affinché il mondo intero sappia di chi stiamo parlando.

con La Fenice e con Trieste, sostenendo che vi è la volontà di risparmio. Ma vi sono situazioni in cui è impossibile risparmiare a causa della struttura stessa. L'Arena è un teatro in cui i padroni pagano da padroni nella platea

una possibilità di investimento che dà molto indotto, come ho già detto, e non voglio ripetermi anche per risparmiare tempo. Chieda agli albergatori, ai ristoratori,

Quest'anno si incomincerà con la "Turandot": meno male che finalmente si inizia con un'opera che non finisce tragicamente, mentre purtroppo, per questo decreto, la conclusione che vediamo avvicinarsi è tragica.

gli emendamenti della Lega avessero solo un impatto mediatico visto che tutti vengono ritirati nonostante la nostra disponibilità. In estrema sintesi, possiamo dire che facevano finta.

dell'articolo 2 è illegittimo, per violazione del principio affermato nell'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, in totale difformità dal Libro V, Titolo 1, Capo terzo, del codice civile. Vorrei che questo rimanesse agli atti, perché è qualcosa che potrà essere oggetto

ha determinato: mi riferisco all'età pensionabile dei ballerini. Il decreto allinea l'età pensionabile a 45 anni sia per gli uomini che per le donne;

per l'età pensionabile massima per i ballerini e i 47 anni per le ballerine, non bisogna andare avanti con la scure, perché rischieremmo di avere dei pensionati a 700-800 euro al mese.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 3.65 (testo 2) e 3.154 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di semplice contrarietà. Resta sospeso il parere sulla proposta 7.0.6 (testo 2)».

probabilmente per un errore di stampa o di grafica, è sempre stata indicata, a partire dall'emendamento 3.338

Signor Presidente, chiedo anzitutto di apporre la mia firma all'emendamento 3.5, presentato dai colleghi Bugnano e Giambrone. L'emendamento è volto alla soppressione del comma 1 dell'articolo il quale prevede che le attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico svolte dal personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche debbano necessariamente essere autorizzate dal sovrintendente, a patto che non pregiudichino le esigenze produttive della fondazione, e devono comunque svolgersi nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale Inoltre, in attesa della sottoscrizione del più volte citato nuovo contratto collettivo nazionale, il presente decreto dispone il divieto ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo sino al 1° gennaio 2011. Invito i colleghi a sostenere con voto favorevole il nostro emendamento, al fine di garantire davvero maggiore autonomia di scelta da parte dei lavoratori.

il Governo su gran parte del provvedimento. Portare la contrattazione di tutto il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche a livello centralizzato mortificare il ruolo dei dipendenti, del personale, delle fondazioni e delle autonomie locali, nonché il ruolo di professionisti di grande validità e competenza.

le prestazioni di lavoro autonomo di personale di grande competenza non mi sembra consono ad un Governo che si autodefinisce ogni giorno con l'aggettivo liberale. *(Applausi

rappresenta un po' il cuore del provvedimento stesso, nel senso che - come ha già detto poc'anzi il collega Rusconi

In particolare, vi è una taglieggio assolutamente crudele dei contratti integrativi che sostanzialmente poi sono la vita reale

Presidente, a conferma di quanto già detto dal senatore Vita, su questo passaggio importante del comma 4 avevamo fatto una riflessione importante in Commissione, che il senatore Asciutti,

noi ci abbiamo creduto, e tutti insieme in Commissione abbiamo stabilito che era opportuno convenire sul 5 per cento perché riteniamo sbagliata e dannosa per i lavoratori quella

ci dica se possiamo accantonare questo emendamento, ci dica se è disponibile a trovare risorse; altrimenti saremo costretti a votare ugualmente l'emendamento, ma si assuma per intero la sua responsabilità davanti ai lavoratori del mondo dello spettacolo.

Poc'anzi abbiamo votato un emendamento della Commissione che portava da uno a due anni il termine per arrivare ad un contratto collettivo nazionale:

In che mondo viviamo se questo Parlamento e la sinistra vanno a difendere le posizioni di privilegio? Questo vi chiedo!

non capisco l'atteggiamento del relatore, che è venuto in Aula a sostenere esattamente l'opposto di quello che è stato sostenuto in Commissione, perché la proposta dell'emendamento 3.47 proveniva dal relatore con l'accordo del Governo *(Applausi dal Gruppo PD).* Credo che sia una vergogna che il Governo non si faccia carico a pieno della responsabilità politica dei provvedimenti che arrivano in Aula, compresa la questione del recupero delle risorse.

ci siamo scontrati, abbiamo trovato dei punti di incontro. Ora, vorrei sapere se queste decisioni le prende il Ministro per i beni e le attività culturali o il Ministro dell'economia

Qual è la *ratio*? Non è una questione tecnica: è una questione di volontà politica! Chiedo al Ministro se è nelle condizioni, credo che lo sia, di far valere la sua volontà. volontà. Siamo di fronte ad un caso in cui il Ministro sostiene che va bene così e poi puntualmente non si è nelle condizioni di far rispettare la propria volontà. Questo è il punto politico che volevo

Signor presidente, onorevoli senatori, non voglio sottrarmi ad un confronto che, nonostante tutto, procede in maniera costruttiva. Su questo punto specifico comprendo le ragioni dei senatori che sono intervenuti, in modo particolare dell'opposizione, ma non solo.

nel caso non si addivenisse entro due anni ad un accordo con riferimento alla contrattazione nazionale collettiva.

da essere intesa in maniera così negativa; semmai, è un incentivo positivo a fare in modo che entro due anni si arrivi al contratto nazionale.

che mi sembra invece molto restrittivo e che finisce per salvare semplicemente al teatro alla Scala. Pensiamo che altre fondazioni meritino di avere la possibilità anche di assumere, se è il caso, e di mantenere alta la qualità delle loro prestazioni.

Presidente, con l'emendamento 3.91 chiediamo che non venga applicata la misura penalizzante del blocco del *turn over* alle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, per alcuni teatri importanti ed, in particolare, per il San Carlo che ha avviato una virtuosa gestione commissariale, alla fine della quale ha risanato la situazione patrimoniale, così come richiesto. Non ho capito bene l'invito al ritiro;

senso appassionato che ha ispirato l'intervento di molti colleghi in questa Aula, come e quanto il Teatro Petruzzelli abbia concorso nel segnare l'identità del nostro territorio e la stessa identità del nostro Paese su un versante così rilevante. Si tratta di un'attività che si è svolta anche attraverso la presenza in questo teatro dei più grandi artisti nazionali e internazionali, che hanno rilanciato in Italia e nel mondo la storia di uno dei più prestigiosi teatri italiani.

ferita lacerante e profonda, non soltanto alla storia di una città e di una Regione ma dell'intero Paese. La specificità e la peculiarità risiedono nel fatto che solo pochi mesi fa, il 4 ottobre, il Teatro Petruzzelli è stato riconsegnato alla pubblica fruizione, visitato dalle più alte cariche dello Stato e ricordo, signor Presidente, che recentemente anche apprezzato come il Teatro sia stato restituito nella sua integrità alla sua funzione fondamentale di organo che propone e promuove cultura ed aggregazione sociale. Questo emendamento ha quindi tre finalità: la prima, prevedere una deroga per quanto attiene le previsioni del comma 5 in ordine all'adeguamento dell'organico; la seconda, che le procedure di assunzione per l'adeguamento dell'organico seguano l'evidenza pubblica; la terza, la previsione di apposite risorse finanziarie, adeguate per la copertura dei costi.

3.154, che rappresenta senz'altro un sostanziale passo in avanti per la soluzione di un problema che affliggeva ed affligge non soltanto la comunità locale, ma anche coloro i quali a livello istituzionale si adoperano perché l'attività del teatro Petruzzelli prosegua. Per queste motivazioni, desidero anche ringraziare il ministro Bondi

per preservare lo sviluppo della storia del nostro teatro e per la garanzia dei suoi operatori.

all'emendamento presentato dalla Commissione e a quelli proposti da me come primo firmatario insieme ad altri colleghi. Vorrei che in quest'Aula ci si assumesse fino in fondo la responsabilità di una chiarezza di posizione, perché se non si è nelle condizioni di esprimersi al meglio per un problema grave, che esiste, bisogna assumersi la responsabilità delle scelte che si fanno, e non contrabbandare interessi e disponibilità e poi ritirare l'emendamento. a queste contraddizioni palesi, non vogliamo tacere: vogliamo mettere in evidenza la difficoltà della maggioranza ad affrontare e risolvere in modo efficace problemi di cui pure è consapevole.

in Commissione il relatore, constatando le discrasie di natura giuridica, si era impegnato a riscrivere il comma 6 dell'articolo 3. Conferma, senatore Asciutti?

è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico-produttivo-organizzativo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro. Dopo aver detto che questo comma non deve essere preso in considerazione, si sostiene esattamente il contrario, vale a dire che deve essere espressamente indicata la ragione per cui si assume a tempo indeterminato. il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non fa altro che attuare la direttiva n. 70 del 1999 dell'Unione europea

abbiano più autonomia e più libertà di assunzione e dunque non si applichino le disposizioni restrittive per quelle fondazioni lirico-sinfoniche che hanno i bilanci a posto. Ci sembra di venire incontro a quanto ieri il ministro Bondi ha affermato in quest'Aula.

Mi associo alle motivazioni esposte dal collega Tofani in relazione all'anticipo del pensionamento dei ballerini.

l'attività lavorativa. Dall'altra parte, poiché stiamo parlando di una ricchezza del Paese, si

brevemente solo per ringraziare il Governo e la Commissione per questo emendamento, che è il risultato possibile

Signor Presidente, si tratta di una questione particolare che è stata sottoposta al Ministro, il quale fin dal primo momento - gliene devo dare atto - si è detto disponibile a considerarla con particolare attenzione.

Noi abbiamo votato e voteremo a favore di questo emendamento come male minore, perché esso non risolve assolutamente il problema del Petruzzelli. Infatti, la deroga che viene concessa è soltanto sulla

uno dei criteri fondamentali per la quantificazione del contributo che lo Stato deve trasferire alle fondazioni conterà moltissimo la qualità della produzione. Ora, se con i fondi ordinari il Petruzzelli non solo deve meritarsi un buon giudizio sul prodotto, che comunque è costoso,

Il Teatro Massimo di Palermo è stato riaperto dopo anni di incuria e mala politica dalla maggioranza di centrosinistra alla fine degli anni '90...

della lirica nel Mediterraneo, un'orchestra, un coro, un balletto di prim'ordine che, con tanti tecnici e maestranze, rappresentano l'eccellenza nell'arte dell'isola, con presenze nazionali ed internazionali.

dalla CONSOB del signor Cardia, su diretto mandato del signor Profumo e di UniCredit, per manipolazione dei mercati. Ero stato accusato insieme all'ADUSBEF di aver provocato il crollo del titolo UniCredit solo per aver denunciato a 10 procure della Repubblica i derivati avariati appioppati dal signor Profumo ad alcune imprese, addirittura portate al fallimento, come la Divania di Bari che dava lavoro a 900 dipendenti. Denunciai subito questo tentativo del signor Cardia (il cui figlio è al libro paga di numerose aziende quotate, vigilate dalla CONSOB) di portare discredito ad un senatore della Repubblica che aveva l'unica colpa di battersi contro le malefatte dell'oligarchia finanziaria e bancaria, di una cricca di potere.

ha annullato quella strana sanzione inflitta per vera e propria rappresaglia. A parte la giustizia penale che farà il suo corso, dal momento che sono iscritti nel registro degli indagati della procura di Roma

di una CONSOB che, invece di sanzionare i comportamenti dei banchieri che hanno prodotto con i derivati e con i CDS miseria e povertà, se la prende con chi difende i diritti dei risparmiatori e dei consumatori. Concludo, signor Presidente, facendo notare che i derivati avariati

a partire dal senatore Rizzi della Lega Nord, ma molti altri sono seguiti (fra gli altri, la senatrice Della Monica e il senatore Ignazio Marino, che addirittura ha segnalato la chiusura degli uffici della Commissione d'inchiesta alle ore 18,30 del venerdì). ci ha rassicurato dicendo che avrebbe fatto le opportune verifiche e ci avrebbe informato sulle decisioni. Quindi, ho chiesto di intervenire semplicemente per essere aggiornata sulle disposizioni

Signor Presidente, intervengo semplicemente per manifestare la mia personale soddisfazione per la sentenza che ha visto assolto il senatore Lannutti

dei termini coloriti utilizzati per raccontare alcuni episodi relativi alla CONSOB, fa sì comunque che la nostra attenzione debba essere alta rispetto ad un organismo di vigilanza

Signor Presidente, colleghi, prendiamo atto con soddisfazione dell'esito favorevole della vicenda che ha riguardato il senatore Lannutti. Pur tuttavia, riteniamo che un inconveniente possa capitare ad ognuno di noi e se, al limite, la CONSOB ha adottato un certo provvedimento, ciò è accaduto in funzione di comportamenti stimolati e che tendevano ad accertare la verità. La verità è emersa. Siamo contenti

posto che universalmente è stato riconosciuto che se in Italia non si sono avuti i guasti registrati in altri mercati europei, lo si deve anche alla competenza, alla diligenza alla vigilanza Per quanto poi riguarda i familiari di ognuno di noi, evidentemente non è fatto divieto che mio figlio eserciti la professione di dottore commercialista, e non per questo gli si possono fare addebiti di sorta, posto che egli esercita questa sua attività nel rispetto delle leggi dello Stato e delle regole della deontologia professionale.